L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo in ordine alle politiche per la riduzione del disagio abitativo.

credo sia stato un atto di grande sensibilità e lealtà da parte del Governo e del ministro Ferrero venire ieri pomeriggio in Aula a riprendere il filo del ragionamento nel merito di un provvedimento molto atteso e peraltro socialmente significativo che riguarda la tutela del diritto alla casa per una fascia debole della popolazione

sempre ribadito, ma mai concretizzato in un provvedimento - della garanzia del trasferimento da casa a casa.

e la necessità dell'opposizione di cogliere l'occasione di

sollevata, alimentata e in qualche modo legittimata da un voto della Commissione bilancio, che per molti versi

venuto a dire in quella sede che vi sono problemi di copertura di un provvedimento che è stato presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro delle infrastrutture.

provvedimenti, che vengono presentati quasi con l'obiettivo di essere affondati. Voglio dire la Commissione bilancio ha alzato una palla talmente bella che l'opposizione avrebbe fatto un errore gravissimo a non coglierla e a non schiacciarla contro il Governo.

che abbiamo il dovere, entro il 29 novembre, di assicurare a queste famiglie una condizione di garanzia,

decaduto aveva il pregio di avviare un piano per l'edilizia residenziale pubblica, un piano per la casa. Ieri il senatore Andreotti ricordava come la politica della casa, a partire dal piano Fanfani, sia stata una delle costanti, cioè lo Stato si è preoccupato di garantire alle fasce più deboli, ai lavoratori, ai cittadini in condizioni di indigenza, il diritto alla casa, il diritto costituzionale all'abitazione. Voglio ricordare che c'era alla base di questo anche uno strumento,

ovvero uno strumento finanziario che aveva anche una funzione per certi versi redistributiva e solidaristica, che finanziava i piani di edilizia residenziale pubblica, la gestione per le case ai lavoratori.

pregherei i colleghi di prendere posto perché è difficile per il senatore Bonadonna intervenire, c'è un brusìo inaccettabile. *(Brusìo)*. Colleghi senatori, pregherei di abbassare il tono della voce, altrimenti è impossibile parlare in questo contesto.

senatore Martone, sottosegretario Vernetti.

politico e politicista, l'attenzione dell'Assemblea cala. Dicevo, improvvidamente è stata cancellata la GESCAL e nel 1992 sono stati sostanzialmente distribuiti i suoi fondi alle Regioni. Il fatto è che questo Paese, oltre ad avere il 4 per cento di edilizia residenziale pubblica contro il 16 per cento della media europea (come ricordava anche ieri il Ministro), si trova da ben quindici anni a non avere alcun finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica. Questo rappresenta un elemento gravissimo su cui bisogna intervenire. Nell'esposizione fatta ieri dal ministro Ferrero si propone un percorso: percorso: il Governo sta studiando la possibilità di produrre un nuovo decreto, cosa che ritengo e che riteniamo assolutamente possibile perché

quindi lo strumento del decreto a nostro avviso può essere utilizzato e, se ho capito bene, grazie alla sensibilità dimostrata anche da interventi che sono venuti ieri dall'opposizione (mi riferisco in modo particolare all'intervento del presidente Matteoli), anche con una corsia preferenziale accelerata che produca un intervento fattivo entro il 29 novembre, in modo da garantire...

la difesa degli interessi delle società immobiliari, ma mi permetto di dire che non solo queste vengono dopo, ma che anche in questo decreto sarebbero state abbondantemente ristorate dagli sgravi fiscali contemplati per coloro i quali avessero

ho colto alcuni elementi, naturalmente dal suo punto di vista assolutamente comprensibili, che possono così riassumersi: è stato un intervento riduttivo sul valore politico della pregiudiziale di costituzionalità; pochi cenni sul da farsi; e una enfatizzazione degli effetti sociali collegati al blocco di questo provvedimento. Pur comprendendo, naturalmente, le ragioni che le hanno ispirato questo suo modo di porgere la questione all'Aula, devo però dissentire profondamente, perché il voto di ieri ha un notevole valore politico; naturalmente, quando dico «notevole valore politico» non intendo riferirmi a possibili crisi di Governo, a divisioni o ad altro, ma sicuramente il voto di ieri è stato, per usare una formula pugilistica, un *uppercut*, un colpo allo stomaco al Governo, che credo ne abbia fortemente risentito. Vede, signor Ministro, anche la questione delle presenze in Aula va vista nella sua giusta ottica: abbiamo in questo inizio di legislatura, parecchie vicende nelle quali la maggioranza ha prevalso per un voto, in assenza di senatori dell'opposizione per le ragioni più varie, per lo più per ragioni giustificate; eppure, in quei casi noi avremmo potuto accampare queste assenze per sostenere che in quell'ipotesi la maggioranza sarebbe andata sotto e quindi avrebbe dovuto lasciare gli scranni del potere. si contano, non si pesano e i voti o i non voti hanno valore prescindendo dalle ragioni del loro esserci o del loro non esserci. Il dato importante, però, che abbiamo potuto verificare è che ieri vi è stata una flebile mobilitazione dei banchi della maggioranza o probabilmente una debole risposta alla mobilitazione per occupare i banchi della maggioranza. Dico ciò,

alla sua base vi erano ragioni ideologiche ed esso, utilizzando il pericolo degli sfratti esecutivi, cercava di introdurre nel nostro ordinamento una serie di norme punitive per la proprietà e per la proprietà delle abitazioni in particolare. Questa volontà politica, questa scelta ideologica ha determinato le forzature costituzionali che noi abbiamo lamentato, cioè l'estensione praticamente a quasi tutto il territorio nazionale del provvedimento, l'esaltazione, quasi, di valori pauperistici ed antiborghesi contenuti nel provvedimento, certamente la sinistra radicale ha imposto alla maggioranza della quale fa parte. Signor Ministro, sappiamo benissimo che questo decreto‑legge fa parte del pacchetto del pacchetto preteso dalla sinistra radicale, magari per ingoiare qualche altro rospo da parte della maggioranza della quale è costitutiva e parte fondamentale.

cioè del patrimonio pubblico acquisito dalle società che hanno partecipato a queste operazioni, e che è dettato, non da ragioni ragioni funzionali alla tutela delle famiglie disagiate, ma da ragioni puramente ideologiche. Si è voluto infatti quasi punire chi ha osato acquisire, a prezzi di mercato, il patrimonio pubblico per metterlo a disposizione della collettività. Signor Ministro, colleghi, questo è un provvedimento che guarda al passato

di quest'epoca: è una visione ottocentesca, o della prima metà del Novecento. Questa visione è però fatta propria da una parte fondante della maggioranza, cioè dalla sinistra radicale, dimenticando che in questi anni vi sono stati un *boom* dell'edilizia e, soprattutto, una diffusione della proprietà immobiliare grazie alla quale grazie alla quale i problemi sociali sono enormemente diminuiti; non dico che non ve ne siano più, ma, ripeto, sono enormemente diminuiti. Questo è un dato di fatto: quasi il 90 per cento delle famiglie italiane è proprietario della casa nella quale abita e questo è un dato che non possiamo assolutamente dimenticare. Ogni azione diretta contro la proprietà degli immobili e in particolare dell'abitazione, è pertanto un'azione socialmente negativa perché colpisce tutti e soprattutto, in questo caso, le famiglie capitolo è cosa fare per il futuro. Noi non vogliamo naturalmente sminuire l'importanza soprattutto della prima parte del provvedimento,

per venire incontro a queste situazioni di disagio. È però chiaro che il prosieguo, nelle Aule parlamentari, dell'*iter* di un provvedimento analogo a quello

Noi - ripeto - non siamo contrari ad un provvedimento a favore delle famiglie disagiate, ma vogliamo che il provvedimento sia rigoroso e, quindi, rispettoso alla lettera dei precetti contenuti nella Costituzione e sviluppati dalla Corte costituzionale; vogliamo che sia funzionale a risolvere quei problemi, vogliamo cioè che non vi siamo ampliamenti nel provvedimento che siano punitivi per la proprietà immobiliare. quindi anche verificare quali e quante situazioni di disagio sono presenti nel nostro territorio. Ho ascoltato ieri l'intervento del Presidente del Gruppo dell'Ulivo, che ha parlato di milioni di famiglie; il Ministro ci parla di 600.000; altri dati ci parlano di 40.000-50.000 casi. Vorremmo sapere con una certa esattezza quali sono i casi ai quali occorre provvedere. Infine, dev'essere un provvedimento equilibrato, che non sacrifichi le famiglie, i proprietari di immobili che si trovino costretti a vedere il rapporto di locazione prolungato nel tempo, ma che vada a carico della fiscalità generale, di tutti e non a carico della fiscalità relativa alla sola proprietà immobiliare. il precetto della Corte costituzionale per cui non si può scaricare sul proprietario l'onere della funzione sociale, in questo caso, della proprietà, sarebbe disatteso; alla fine sarebbe sempre la proprietà immobiliare a pagare le conseguenze: devono pagarle, invece, tutti i cittadini. Annuncio anche che Forza Italia ha presentato ieri un disegno di legge a prima firma del senatore Schifani in questa direzione, un provvedimento rigoroso, funzionale ed equilibrato.

Signor Presidente, il ministro Ferrero ha enunciato le preoccupazioni del Governo, che il Gruppo dell'Ulivo condivide, in ordine alla bocciatura del decreto-legge in materia di disagio abitativo. Ha anche indicato una via possibile per introdurre nuove norme in tema di edilizia abitativa, norme che dovranno guardare - noi ci auguriamo - oltre l'emergenza, puntando sulla prospettiva dei piani di edilizia residenziale pubblica ed anche su misure equitative a favore dei conduttori deboli. In questo quadro, credo che si dovrà intervenire con una misura a tempo sulle situazioni di particolare disagio, che sono quelle nelle quali è in corso una procedura di sfratto nei confronti di persone e famiglie appartenenti alle categorie più disagiate e alle fasce sociali più deboli. Ci accingevamo ieri ad affrontare i singoli problemi posti da questa normativa e, tra l'altro, a sciogliere le questioni che erano state sollevate dalla 5a Commissione con i suoi pareri: sfavorevoli a due degli emendamenti e favorevoli ad un emendamento soppressivo del comma 7 dell'articolo 1. pausa di riflessione che avevo chiesto non c'è stata, il Governo si apprestava a presentare emendamenti che avrebbero reso necessaria la fissazione di un termine per eventuali subemendamenti. In quel momento, dopo le nostre relazioni, la scelta dell'opposizione nel suo insieme è stata quella di puntare sull'approvazione di una pregiudiziale tale da far colare a picco l'insieme del decreto-legge. Avremmo potuto risolvere secondo le procedure parlamentari le questioni relative alla copertura di quelle norme e attendevamo la proposta del Governo su questo tema. Invece no: no: approfittando di una situazione nella quale vi era una temporanea lieve maggioranza a favore delle forze di opposizione, la scelta che avete compiuto è stata di liquidare nel loro insieme queste norme. Voglio rispondere alle questioni poste ieri dal collega Matteoli (che non vedo nei banchi di Alleanza Nazionale), il quale ha sollevato quesiti ai quali è necessario, da parte nostra, fornire una risposta. Il senatore Matteoli ha chiesto se il Governo ha una maggioranza. Ebbene, parliamoci chiaro: voi sapete quali sono i rapporti di forza dentro quest'Aula e come sia ristretto il margine del quale possiamo disporre. Tuttavia, vorrei serenamente rispondere al collega Matteoli: sì, il Governo ha una maggioranza e lo ha dimostrato in un voto politico, qual era quello di ieri pomeriggio sulle dimissioni di uno dei nostri colleghi che fanno parte del Governo; lo ha dimostrato a voto segreto di avere una maggioranza. Naturalmente, il percorso di approvazione di norme delicate e oggetto di discussione è sempre accidentato. Capiterà che voi riusciate,

Potevate aspettare le votazioni su quegli emendamenti soppressivi, tra l'altro assistiti dal parere favorevole della 5a Commissione, per far valere il vostro punto di vista.

Mi fa piacere sollecitare qualche reazione, invece che parlare nella disattenzione generale. Le reazioni sono benvenute. *(Commenti del

appellandomi alla vostra attenzione, io formulassi un giudizio di valore sulle posizioni o sulla cultura dell'una o dell'altra forza politica. Vede, collega Matteoli, l'atteggiamento da tenere, a mio giudizio, nei nostri dibattiti e nella lotta politica di cui noi siamo parte e protagonisti, dev'essere sempre improntato al rispetto nei confronti degli avversari. Rispettare gli avversari significa anche, in qualche misura, rispettare sé stessi. Allora, nel pieno rispetto delle vostre posizioni io mi sono limitato ad osservare, e ancora oggi su questo richiamo la vostra attenzione, che le famiglie colpite dall'affossamento del decreto sono le famiglie dei ceti popolari, la gente delle periferie. Siccome i vostri partiti prendono un certo numero di voti

*(Applausi dal Gruppo Ulivo)*. Invece, per una scelta di schieramento voi affossate il decreto rendendo impossibile in questo momento una proroga congrua della sospensione degli sfratti. Questo è il dato politico! Questo è il rilievo della scelta compiuta ieri da voi approfittando della posizione di vantaggio in cui vi trovavate! Il Governo ha assunto degli impegni la maggioranza farà tutto quel che può affinché norme nuove che corrispondano agli interessi, alle esigenze, ai diritti di quelle persone, di quelle famiglie siano varate quanto prima dal Parlamento italiano. Voglio rassicurare il collega D'Onofrio: non è in discussione il diritto di proprietà. In quelle norme equilibrate ieri in discussione era perfino recepito dalla giurisprudenza costituzionale il principio della comparazione tra la posizione del locatore e la posizione del conduttore. Certo, vi erano maggiori garanzie per i conduttori deboli quando la parte locatrice era una grande proprietà; ma questo corrisponde all'articolo 3 della Costituzione repubblicana ed anche all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione repubblicana. Il collega D'Onofrio lo sa bene. Non vi era scontro ideologico su quelle norme e avremmo potuto comunque trovare un'intesa, anche accogliendo esigenze ed emendamenti da voi posti, come, del resto in Commissione avevamo accolto all'unanimità l'emendamento proposto dal collega Caruso. Avete voluto la rottura per ragioni politiche e di schieramento e di questa scelta dovrete rispondere all'elettorato! Essendo terminati tutti gli interventi nella discussione sulle comunicazioni del Governo in ordine alle politiche per la riduzione del disagio abitativo, passerei al prossimo punto all'ordine del giorno.

La questione che pongo è la seguente: è prevista o meno la replica del rappresentante del Governo? Lo chiedo per un motivo molto semplice. Ho apprezzato la disponibilità del Ministro per arrivare ad una strada possibilmente condivisa; poi se ci arriveremo si vedrà. Vedo però da parte del Capogruppo del maggior Gruppo di maggioranza

mediante procedimento elettronico, sulle dimissioni presentate dal senatore Pinza. I senatori favorevoli ad accogliere le dimissioni premeranno il tasto verde al centro della postazione di voto; i senatori contrari premeranno il tasto rosso a destra; i senatori che intendono astenersi premeranno il tasto bianco a sinistra. Poiché si tratta di uno scrutinio segreto, qualunque sia la scelta di voto effettuata, la luce che si accenderà sarà di colore neutro.

di procedere all'accertamento del candidato subentrato ai senatori dimissionari, autorizzo la Giunta a convocarsi fin d'ora. Passiamo Passiamo al prossimo punto

se la seduta viene sospesa o meno per consentire alla Giunta delle elezioni di lavorare, perché ieri il presidente Marini ha agito secondo questa procedura. Questo prescinde dal fatto che l'Aula voti o meno perché chiunque tra noi potrebbe ora presentare chiunque tra noi potrebbe ora presentare una sospensiva o qualunque questione che lei non è in grado di prevedere. L'Aula va sospesa e fra dieci minuti, quando la Giunta ha finito, si riprende. Non credo che sia possibile fare in maniera difforme rispetto a ieri.

i nostri lavori. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Emilia-Romagna, a seguito delle dimissioni del senatore Roberto Pinza, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Luca Marcora.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

una nuova finestra") *(AN)*. Signor Presidente, Ministro, onorevoli colleghi, quello che si è finora fatto in materia di immigrazione esprime in modo paradigmatico la politica di questo Governo, irresponsabile, improvvisata, superficialmente demagogica. L'annuncio ripetuto di sostanziali sanatorie e di regolarizzazioni, la proposta del Ministro dell'interno che gli immigrati clandestini ricevano dallo Stato soldi per tornare nel loro Paese, la regolarizzazione di quei clandestini che denuncino i datori di lavoro, l'indebolimento (che è premessa di un sostanziale smantellamento) dei Centri di permanenza temporanea, la promessa della concessione di una cittadinanza abbreviata e la previsione di ampi ricongiungimenti parentali che vanno ben al di là del nucleo familiare hanno determinato un effetto-richiamo che ha già prodotto risultati impressionanti con un aumento vertiginoso degli sbarchi. Mi sembra oggettivamente irresponsabile, anche per la sua sostanziale legittimazione di una grave illegalità, la proposta del Ministro dell'interno di dare soldi ai clandestini per incoraggiarli a rientrare in patria. Mi chiedo come non accorgersi del circolo perverso che si innescherebbe!

allora, si diano i soldi alle forze dell'ordine, si facciano finalmente le espulsioni e si costruiscano i Centri di permanenza temporanea. Devo sottolineare a questo proposito che in finanziaria purtroppo non c'è nulla in materia di sicurezza, non c'è nulla per le forze dell'ordine. Per venire specificamente al cosiddetto decreto flussi, la sua gravità è rappresentata da una serie di elementi. Esso stravolge il significato stesso di un decreto di programmazione dei flussi che serve - appunto - a programmare gli ingressi e non a sanare forme di clandestinità: voi, infatti, state facendo una sanatoria.

le organizzazioni sindacali hanno coerentemente proposto per questi stranieri l'esenzione dal visto di ingresso. Nona caso, dunque, il decreto prevede 350.000 nuovi permessi che si vanno ad aggiungere ai 170.000 già programmati e che rappresentano la differenza rispetto al totale

C'è il rischio che il nostro Paese si riempia di persone senza stabile occupazione che potrebbero saldarsi con quei 10.000 extracomunitari che l'indulto ha improvvidamente liberato senza garantirne l'espulsione e che, come risulta dalle cronache, in buona parte sono tornati a delinquere. C'è il rischio che, anziché essere noi a trasmettere la nostra identità, si dia vita ad una società senza identità e senza valori di riferimento. Si tratta dunque di una sanatoria che si vuole mascherare di fronte all'opinione pubblica e all'Unione Europea, dato che ogni provvedimento di sanatoria ha bisogno di un accordo con la Commissione europea. europea. Forse è più grave il fatto che per raggiungere lo scopo si arriva ad aggirare la legge e si propone un *escamotage* che solo chi ha un basso senso di legalità e del diritto può immaginare: si finge che la domanda sia stata presentata da chi sta all'estero, mentre si tratta di un clandestino già presente in Italia. Esemplari sono al riguardo le parole del Ministro dell'interno! Dunque, si chiede implicitamente alle nostre autorità di frontiera di chiudere gli occhi perché la legge prevede invece che, quando il clandestino esce dalla frontiera, l'autorità di polizia debba contestargli l'irregolarità dell'ingresso e notificargli con l'espulsione il divieto di ingresso per i successivi dieci anni. Insomma, si auspica la commissione di un reato da parte della Polizia di frontiera; viene meno il collegamento con il contratto di lavoro, come fissato invece fin dal giugno 2002 dal Consiglio europeo di Siviglia; in sostanza, passa la linea più radicale per cui l'Italia deve diventare una sorta di terra aperta a chiunque, a prescindere dalla possibilità di integrazione e dalla necessità del nostro sistema produttivo. è esattamente il contrario di quanto serve ad una politica delle integrazioni. Voi create le premesse per la nascita di sacche esplosive di disagio, di emarginazione e di potenziale illegalità. In poche parole, state creando le premesse per la disgregazione del nostro Paese: ogni giorno che passa fornite una prova in più della vostra incapacità ad esprimere un'azione di Governo avveduta e responsabile nell'interesse della nostra Nazione.

Signor Presidente, l'immigrazione è un nuovo, grande e profondo fenomeno sociale del XXI secolo. Non si tratta oramai di un fenomeno contingente, ma di un aspetto strutturale della società italiana. Lo è, prima di tutto, per fattori demografici: la forte depressione della natalità sta trasferendosi rapidamente sulle giovani leve della popolazione attiva, che sono in forte diminuzione. Lo è perché una parte rilevante del sistema produttivo dei beni e dei servizi è costituito da attività ad alta intensità di manodopera, che di frequente non è reperibile tra i nostri connazionali. Lo è, infine, perché un sistema di *welfare* assai arcigno verso le famiglie rende conflittuali le funzioni di allevamento e di cura dei figli con l'impegno nel mercato del lavoro o con l'attività di cura e sostegno degli anziani non autosufficienti, che crescono rapidamente di numero: viene così esaltata una domanda di lavoro domestico che non ha eguali in Europa. La normativa attualmente in vigore per l'ammissione di immigrati per lavoro è assai inefficiente, perché apre quasi esclusivamente una sola via di accesso al lavoro nel nostro Paese: la cosiddetta chiamata diretta o numerica del cittadino estero da parte del datore di lavoro che quasi sempre tale cittadino non conosce. E' un sistema inefficiente, per le famiglie come per molti altri datori di lavoro, che hanno necessità di un incontro diretto con l'immigrato prima di deciderne l'assunzione. Avviene così che gli stranieri non comunitari arrivino, per lo più regolarmente, cerchino e trovino un lavoro generalmente al nero, e si convertano così in irregolari. Questa bolla di irregolarità tende ad espandersi rendendo inevitabile il suo «svuotamento» periodico attraverso le sanatorie, l'ultima delle quali, nel 2002, regolarizzò la posizione di oltre 700.000 lavoratori. In altra mozione si solleva il dubbio che il decreto integrativo sui flussi per l'anno 2006 altro non sia che una sanatoria mascherata di quegli irregolari che non sono rientrati tra i 170.000 previsti dal primo decreto Berlusconi e che ad essi pertanto dovrebbe applicarsi un decreto di espulsione con divieto di riammissione in Italia. Ma perché mai questo dovrebbe valere per gli immigrati dal centosettantamillesimo posto in poi tra quelli che fecero domanda il 14 marzo scorso e non per i primi 170.000 rientrati nel decreto Berlusconi? Per quale ragione, o miracolo, domande presentate contemporaneamente dovrebbero riferirsi a due categorie diverse di persone, nettamente divise da tale fatidico numero d'ordine? La normativa vigente, inoltre, prevedendo permessi di soggiorno di breve durata e di laborioso e difficile rinnovo - il che crea un limbo nei diritti dell'immigrato regolare nelle more del rinnovo stesso - è inutilmente vessatoria per gli ospiti stranieri ed onerosa per l'amministrazione. Anche su questa materia è urgente

dannoso, costoso quanto inefficiente di irregolarità, espulsione ed arresto, criminalizzando l'intero fenomeno e gettando un'ombra sulla maggior parte degli immigrati che vogliono pacificamente integrarsi nel nostro Paese. Infine, i processi di integrazione sono stati colpevolmente trascurati dal passato Governo: ne fanno testimonianza la soppressione del Fondo per l'integrazione ed il mancato rinnovo della commissione per l'integrazione, ambedue previsti dal vigente testo unico. Ma un Paese nel quale l'immigrazione è una necessità strutturale ha bisogno di potenti sostegni ai processi d'integrazione: casa, formazione, cultura e scuola. Il binomio immigrazione-integrazione è inscindibile e va al più presto ripristinato. Queste brevi considerazioni rendono evidente l'urgenza e la rilevanza dell'impegno del Governo nel complesso campo dell'immigrazione. Fermo restando il principio non negoziabile della difesa della legalità e del contrasto all'irregolarità nel pieno rispetto dei diritti civili, l'azione deve procedere lungo alcune fondamentali linee. programmazione realistica dei flussi, basata su indagini oggettive ed approfondite, possibili ma fino ad oggi assenti. In secondo luogo, pluralità delle vie d'accesso legali per rendere possibile l'incontro tra domanda ed offerta, circoscrivendo il fenomeno dell'irregolarità; questa può essere anche ridotta, non solo con politiche coercitive e repressive ma anche con incentivi e forme premiali. In terzo luogo, concessione di permessi di soggiorno per periodi più lunghi e meccanismi di rinnovo non vessatori per gli immigrati ed onerosi per l'amministrazione. luogo, costruzione di politiche dell'integrazione provviste di adeguate risorse e seriamente monitorate per le prime e, soprattutto, per le seconde e le terze generazioni; conclusione della riforma dei processi di acquisizione di cittadinanza risibilmente rari, oggi, nei confronti delle esperienze degli altri Paesi europei. Infine, rafforzamento delle politiche bilaterali e multilaterali con i Paesi d'origine che ponga i processi migratori al centro delle nostre politiche di sviluppo. Le migrazioni vanno governate e incanalate nelle vie legali, nell'interesse delle società di partenza e di quelle di destinazione. Colleghe e colleghi del Senato, l'immigrazione è parte viva del nostro Paese: sostiene lo sviluppo, protegge il nostro benessere e determina importanti mutamenti sociali. Va però governata, come un fenomeno di lungo, lunghissimo periodo, al di sopra e al di là delle polemiche, dei calcoli e delle convenienze contingenti.

illustrerò velocemente la mozione proposta dal nostro Gruppo, che ovviamente vuole richiamare il Governo a ritornare sui propri passi, soprattutto per quanto riguarda il provvedimento relativo all'ampliamento ad ulteriori 350.000 cittadini extracomunitari della quota di flusso prevista per il 2006. Richiameremo il Governo ad un comportamento più corretto e a non commettere un falso ideologico come sta facendo, chiamando questo momento di flussi semplicemente una sanatoria. L'aumento di flussi, infatti, dovrebbe comunque seguire quanto previsto dalla legge Bossi-Fini, attualmente in vigore, e non diventare sostanzialmente - come dichiarato da più Ministri - una sanatoria per 350.000 cittadini, presenti già nel nostro Paese in maniera irregolare. Ricordo peraltro che, poiché moltissimi di questi cittadini hanno fatto domanda in più sportelli postali, in realtà anche il numero di 350.000 è probabilmente sovrastimato, quindi, oltre a quelli presenti irregolarmente ne chiamerà ulteriormente degli altri. Questo è in sostanziale contrasto con quello che il primo ministro Prodi va dicendo in giro per l'Europa: si incontra con i responsabili francesi, inglesi, con lo spagnolo Zapatero, parlando di sicurezza delle frontiere europee e poi di fatto in Italia fa l'esatto contrario, o perlomeno lo fa fare ai propri Ministri, come il ministro Ferrero. Anche a tal proposito bisognerebbe ricordare proprio il problema legato alla sicurezza e ai costi sociali di questo fenomeno perché qui mi sembra che si sta veramente confondendo la realtà dei fatti e si stanno facendo affermazioni assolutamente inesatte. Ricordo che fino a prima della Bossi-Fini gli extracomunitari iscritti all'INPS erano solo 400.000; con la Bossi-Fini sono diventati circa un milione, con i 600-700.000 regolarizzati, facendoli emergere dal lavoro nero. Quindi oggi, a fronte di 4-5 milioni di extracomunitari presenti nel nostro Paese, ne lavora non più di un milione in regola. Rendetevi conto del tasso di occupazione, metà di quello italiano, che è già bassissimo, e dei costi sociali relativi ai tre cittadini stranieri che non lavorano a fronte di uno solo che lavora normalmente (oltre tutto il lavoro è a basso valore aggiunto); quindi, il vostro modo di affrontare il problema migratorio è l'esatto contrario di quanto previsto dalla Bossi-Fini, che è assolutamente in linea con quanto previsto da tutte le normative europee, cioè una legge legata alla possibilità di lavoro, di abitazione, di inserimento sociale. La vostra politica è quella dei ricongiungimenti facili (ricordiamo i parenti di quarto grado della Turco-Napolitano), un anno per ricerca di lavoro che significa togliere ogni clandestinità, perché evidentemente qualunque cittadino trovato in stato irregolare nel nostro Paese potrà dichiarare che sta ricercando un lavoro e diventa in automatico regolare. Spiegatemi allora come faranno ad esserci in futuro extracomunitari irregolari.

per sostituire nel voto i cittadini italiani vecchi, cioè quelli veri, che ormai, dalla prossima elezione in poi, non vi voteranno più. Lo stesso si può dire per il diritto di sangue sostituito dal diritto di suolo, che è un elemento che stravolge 2.000 anni di storia.

che i cittadini danno alla Lega Nord per l'indipendenza della Padania: questa si chiama pulizia etnica elettorale. Qualche mese fa ho letto un libercolo che mi hanno regalato, che porta il titolo «Mein Kampf», di un autore del secolo scorso, tedesco di origini austriache, che diceva esattamente le stesse cose; in quel caso la pulizia etnica veniva fatta in maniera un po' diversa, ma il ragionamento era esattamente lo stesso. Finché si scherza, Finché si scherza, finché si parla di soldi, di finanziarie, va bene tutto, perché poi ci penseranno i Governi che verranno dopo, quelli normali, a rimettere in sesto dal punto di vista economico il Paese. Anzi, personalmente ritengo che un paio di vostre finanziarie - perché di più non credo che ne farete - siano quasi positive per il Paese, perché per lo meno i cittadini che vi hanno votato e tutti gli altri si renderanno conto di cosa vuol dire avere i comunisti al potere. Qui però c'è in gioco il futuro del Paese, che è un'altra cosa:

perché gli italiani sono 58 milioni da zero a 100 anni, mentre gli extracomunitari sono 5 milioni mediamente da 15 a 45 anni. Hanno un tasso di sviluppo enormemente superiore al nostro, tant'è che già oggi, a fronte dell'8-9 per cento di extracomunitari, le nascite di bambini figli di extracomunitari sono nell'ordine del 15-20 per cento. Se voi ne fate entrare altri 6.000.000-700.000 all'anno, fra una generazione ci troveremo un Paese con maggioranza extracomunitaria e magari con una forte prevalenza, fra gli extracomunitari,

dice: «Sappiamo benissimo che quelli che hanno fatto la domanda sono già presenti sul nostro territorio e quindi sono irregolari, ma dovremmo rimandarli al nostro Paese per farli tornare indietro? Non fatemi ridere». Abbiamo, quindi, un Ministro dell'interno che ufficialmente afferma che tollera una irregolarità, un reato nel nostro Paese, e dice che va bene così. È lo stesso Ministro rappresentante del Governo che invece, per uno scontrino fiscale, vuole far chiudere i negozi degli italiani e se persona non denuncia una irregolarità presunta può prendere fino a 2.000 euro di multa perché non ha fatto il delatore. Che il ministro Amato possa odiare gli italiani e tutto quello che è occidentale possiamo anche capirlo, che voi possiate andare al 20 per cento dei voti è estremamente probabile, viste le cose che stiamo facendo, ma certo se voi rimarrete qualche anno al Governo sarete in grado di distruggere completamente e irreversibilmente il Paese*.* Al mondo ci sono i comunisti furbi, come Zapatero, che concede il matrimonio ai *gay*, ma poi dà l'indipendenza alla Catalogna, ai baschi, ma soprattutto ha introdotto una

alcuni colleghi intervenuti precedentemente, di una sanatoria mascherata e questo è un fatto estremamente grave. In secondo luogo, il decreto in oggetto esprime una linea di tendenza dell'attuale maggioranza parlamentare

usa metodi molto duri per impedire gli sbarchi alle Canarie e dà il via ad una rilevantissima operazione di espulsione di circa 800.000 clandestini.

che aumenti il fenomeno dell'immigrazione clandestina, in particolare islamica, la quale provoca una rottura sociale nel Paese. Vi è poi Blair che, dopo la vicenda degli attentati di Londra, ha deciso di cambiare completamente politica in Inghilterra, dichiarando finita la politica dell'integrazione multiculturale e dell'integrazione multietnica. Detto da Blair, è un fatto di grande rilevanza perché il modello dell'integrazione multiculturale era il punto di riferimento dell'intera sinistra italiana.

Perché, quando c'è da parlare di diritti civili, la sinistra italiana guarda con grande attenzione a Zapatero, oppure, quando c'è da riferirsi a nuove sperimentazioni del riformismo, guarda con grande attenzione alla "terza via" di Blair, mentre, quando c'è da parlare di gestione, di controllo dell'immigrazione e di governo dei flussi migratori, le politiche che questi due *leader* della sinistra europea adottano non vanno più bene?

di una sinistra radicale che non tiene conto delle compatibilità del Paese e dei pericoli che esso sta correndo con questa politica lassista e di apertura nella gestione dei flussi migratori.

In questo sondaggio appariva con chiarezza che la maggiore preoccupazione, anche dell'elettorato di centro-sinistra o della sinistra moderata, era legata alla questione migratoria e ai problemi della sicurezza.

anche a settori mafiosi, che operano nel nostro Paese e nei Paesi di provenienza e che organizzano l'arrivo delle badanti e la loro distribuzione sul territorio nazionale.

la nostra, di frontiera (che è la vera porta dell'immigrazione clandestina), vede ormai sull'autostrada un passaggio continuo di pullman che arrivano dall'Ucraina, dalla Moldavia e dalla Romania. Dietro questi pullman che portano cittadini o cittadine di quei Paesi, che vorrebbero trovare un lavoro in Italia e che vengono nel nostro il semplice visto di soggiorno turistico, c'è un'organizzazione di interessi e di tratta delle persone su cui non dite niente.

non ha assolutamente detto niente. Provate a pensare ad un'altra struttura che si occupa della gestione di queste persone, cioè le cooperative di servizi, talvolta iscritte alla famosa Lega delle cooperative. Esse utilizzano questa forza lavoro, questa povera gente, speculandovi sopra in modo rilevantissimo. Da parte vostra non si dice niente. Accanto alla gestione

Ieri avete gridato allo scandalo perché è stato bocciato il decreto-legge sugli sfratti, ma non vi preoccupate del fatto che, accanto a quei 10.000 casi di sfratti, ci sono centinaia di migliaia di casi di povera gente che non sa dove andare a dormire e di cui favorite l'ingresso.

il governo dei flussi migratori, che va gestito con serietà, è il vero fenomeno di questi anni che dobbiamo vivere. Non solo la gestione del fenomeno dell'immigrazione dai Paesi islamici, che rischia di creare i fenomeni negativi che si sono avuti nell'Inghilterra di Blair, ma soprattutto il passaggio di questa gente proveniente dai Paesi dell'ex Unione Sovietica rappresenta un altro fenomeno che rischia di incidere profondamente sul nostro tessuto sociale.

gente che proviene da più storie e tradizioni, ma in modo regolato: è possibile lasciare questo processo di immigrazione completamente ingovernato e ingovernabile? Voi rischiate di portare l'Italia al disastro.

e non si cerca di prendere atto soprattutto del fatto che i 10.000 extracomunitari che sono usciti di galera grazie all'indulto dovrebbero essere espulsi per primi, visto che non siete stati in grado, accanto all'indulto, di costruire un sistema di integrazione di questa povera gente. A questo punto, rimettendoli in giro, usciti dalla dalla galera, senza un posto di lavoro, continueranno a delinquere, provocando un altro disastro nell'opinione pubblica del nostro Paese. *(Applausi

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, io sono un comunista anche se spero di non fornire troppi elementi per essere iscritto nella categoria dei cretini, come ha fatto il senatore Galli.

chiedono al Governo di porre in essere una serie di misure, tra cui la revoca del decreto flussi integrativo, tutte restrittive e punitive nei confronti degli immigrati. Tali misure, se se attuate, risulterebbero al limite della costituzionalità e certamente in violazione dei princìpi fondamentali in materia dei diritti umani. Non bisogna dimenticare che la posizione dell'Europa in materia di immigrazione trova un'importante testimonianza nella risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre scorso. In essa si riconosce la necessità di aumentare in in futuro i flussi migratori per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro dell'Unione Europea e per garantire la prosperità dell'Europa;

si afferma la necessità che l'Unione Europea offra possibilità concrete di immigrazione legale; soprattutto, si riconosce la necessità che gli Stati membri possano adottare approcci differenti al problema della presenza di centinaia di migliaia di immigrati clandestini che lavorano illegalmente e senza alcuna protezione sociale.

di ergersi a paladino di un proprio individuato insediamento sociale, dobbiamo insieme cercare di operare per l'interesse generale di questo Paese. Anche le

o, addirittura, ancora cercano lavoro (e sono tanti) la presenza di lavoratori immigrati è un problema interno al mondo del lavoro.

porre al più presto mano alla cancellazione della legge Bossi-Fini; deve scrivere una legge moderna che affronti i problemi non per cercare i voti di quelle componenti moderate del Paese pronte allo scontro con chi è portatore di una cultura diversa. Bisogna vedere l'arricchimento culturale e guardare con simpatia a quei giovani immigrati che, nonostante le enormi difficoltà, riescono

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, intervengo su questo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea perché mi sembra davvero irragionevole ed irresponsabile da parte del Governo intervenire su una problematica così complessa e delicata come la questione riguardante l'immigrazione attraverso provvedimenti frammentati, che creano solo confusione e incertezza. Soprattutto il provvedimento relativo ai flussi migratori assume sempre più le vesti di una vera e propria sanatoria, che viola in modo palese la legge italiana sull'immigrazione, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura, meglio conosciuta come legge Bossi-Fini. In diverse occasioni gli esponenti della maggioranza hanno annunciato di voler modificare la normativa attualmente vigente, ma ad oggi nessun esponente del Governo ha presentato un disegno di legge organico come proposta di modifica del testo unico previsto in materia. L'unico provvedimento - come ho detto - adottato fino ad oggi è il decreto flussi integrativo. Si tratta di uno strumento prettamente di ordine amministrativo che prevede il criterio secondo cui a tante domande presentate devono corrispondere altrettanti ingressi regolari. E questo principio - a nostro avviso - non è accettabile. Ci troviamo in una situazione assurda ed irragionevole, con un Governo che continua a proporre provvedimenti finalizzati unicamente alla distruzione il tutto ciò che è stato fatto dal precedente Esecutivo. Tale strumento di ordine amministrativo, difatti, non fa altro che minare irrimediabilmente l'intera normativa della legge sull'immigrazione; legge che ha fornito una risposta più che soddisfacente al sempre maggiore crescente problema dei clandestini nel nostro territorio. Come dicevo, in molte occasioni il Governo ha palesato la sua volontà di voler modificare la normativa vigente sull'immigrazione, di voler modificare il limite temporale per l'acquisizione della cittadinanza italiana, di voler intervenire sul sempre più frequente fenomeno degli scafisti, ed ancora sulla possibilità del ricongiungimento familiare, con estrema leggerezza ed incoscienza, attraverso uno strumento di puro ordine amministrativo e non rimettendo al Parlamento la decisione tramite il corretto *iter* legislativo.

Difatti, è proprio il Parlamento che deve essere chiamato a decidere, esercitando in tal modo la sua competenza. La maggioranza, invece, temendo una bocciatura di eventuali provvedimenti in merito, preferisce adoperare strumenti più sicuri ma meno corretti, come appunto i decreti interministeriali, espropriando in tal modo l'Aula del Parlamento della sua competenza e limitandosi all'espressione di un semplice parere in Commissione. Onorevoli colleghi, siamo arrivati all'assurdità. Il Governo si vede costretto ad utilizzare strumenti inadatti per ottenere qualche risultato, ma così facendo non si rende conto che non solo si approvano provvedimenti che peggiorano il fenomeno dell'immigrazione, ma si alterano anche quei rapporti e quegli equilibri internazionali raggiunti faticosamente dal precedente Governo attraverso accordi con i Paesi interessati al fenomeno. decreto flussi integrativo il Governo italiano non solo disapplica una legge dello Stato ma, ciò che è ancora più grave, elimina uno dei punti principali della normativa dell'Unione Europea in materia d'immigrazione, ovvero fa venir meno il collegamento tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro sostituendolo con un presupposto completamente diverso, quale la semplice concessione di detto permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari già presenti clandestinamente in Italia. Colleghi, è di questo che si tratta, ed è stato più volte confermato dagli esponenti della maggioranza durante i lavori della Commissione affari costituzionali. Le innumerevoli file per la presentazione della domanda per vedersi riconosciuto il permesso di soggiorno sono state fatte proprio dai diretti interessati, clandestini, a dimostrazione che queste persone sono già presenti nel nostro Paese. La paradossale soluzione a questo problema, prospettata da parte del Governo ed in particolar modo dal ministro Amato, è stata quella di ipotizzare, per i clandestini, il finanziamento per il rimpatrio volontario. Secondo tale proposta, chi dovrebbe essere espulso, anziché essere condotto coattivamente alla frontiera, riceverebbe una somma di denaro per il volontario e libero rientro in patria. Mi chiedo con quale coraggio o con quale ingenuità si possa ipotizzare una simile soluzione! Porre il clandestino in una tale situazione significherebbe legalizzare un circolo vizioso. Difatti, i destinatari di tali somme di denaro non farebbero altro che pagare, con parte del denaro, un falso documento per una nuova identità e ritornare nel nostro territorio fino ad essere nuovamente scoperti e nuovamente riforniti di denaro per l'allontanamento libero e volontario. Onorevoli colleghi, occorre prendere atto della gravità di detti provvedimenti e pretendere dal Governo un impegno maggiore, e soprattutto più ragionevole, su questa delicatissima ed importante materia, per combattere in maniera più efficace il fenomeno dell'immigrazione clandestina che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Quello che chiediamo è che il Governo applichi la già esistente legge in materia di immigrazione e continui a mantenere l'attuale disciplina del ricongiungimento familiare, che ritenga prioritario l'allontanamento effettivo dei clandestini scarcerati dal recente provvedimento di indulto e, soprattutto, che si riprenda un'effettiva e proficua collaborazione con i Paesi di provenienza dei clandestini, sviluppando semmai accordi sempre più efficaci, che introducano nuove norme organiche, che migliorino i punti che si sono rivelati deboli in fase attuativa della legge vigente. L'UDC dà la propria disponibilità ad un voto favorevole, ma su una mozione unitaria, concordata con tutti i Gruppi di opposizione.

Signor Presidente, senatrici e senatori, l'amministrazione comunale di Padova ha avviato l'assegnazione di abitazioni civili, a canoni compatibili, agli immigrati che risiedono negli alloggi fatiscenti di via Anelli. È una decisione da salutare positivamente, dopo le non poche perplessità che la costruzione del muro aveva provocato. Un servizio televisivo della trasmissione «Primo Piano» ci ha informati lunedì sera che questa assegnazione ha fatto registrare vibrate proteste. Era da attendersi che a protestare fossero cittadini che spesso individuano nell'immigrato il capro espiatorio delle proprie insoddisfazioni. Non è stato così. In base all'inchiesta del servizio, le maggiori proteste per questa assegnazione e conseguente trasferimento sono state sollevate dai proprietari di quegli alloggi fatiscenti che erano stati locati agli immigrati ad affitti esorbitanti e, presumibilmente, senza regolare contratto e certificazione; in nero, insomma, come spesso si dice e ancora più spesso si fa in questo Paese. Non è singolare che ciò sia avvenuto. In moltissimi casi la questione degli immigrati viene affrontata da due angolazioni contraddittore: da un lato, si sollevano scandali e preoccupazioni per la nostra sicurezza e per i rischi che correrebbe la nostra identità nazionale; dall'altro, gli immigrati costituiscono fonte di arricchimento illecito nelle attività produttive o nel godimento coatto di servizi al di sotto della soglia della decenza. In moltissimi casi a sollevare lo scandalo e ad usufruire dei vantaggi che derivano dall'immigrato è la stessa persona. A mio parere, questa doppiezza deriva in parte da una concezione della legalità che individua i soggetti da cui pretenderla soltanto, o prevalentemente, negli strati più deboli della popolazione, siano essi cittadini italiani o immigrati. È una concezione diffusa che si fonda sull'impunità dei potenti e dei forti che richiama, purtroppo, tensioni, invidie e tentativi di imitazione a vari livelli e finisce con il produrre corruzione del tessuto civile e morale della società e pericoloso nocumento alla stessa esigenza condivisa di legalità. Nello specifico dell'immigrazione, questa concezione parziale e a senso unico della legalità finisce con il rendere appetibile e conveniente il fenomeno dei clandestini, braccia a bassissimo costo senza il godimento dei diritti più elementari, utili persino per i profitti di gestione di un CPT, cioè di un centro di permanenza più o meno temporanea. Un coraggioso giornalista ce ne ha offerto recentemente ampia prova. Resta da chiedersi se dovremmo avere ancora bisogno di inchieste coraggiose, soprattutto quando leggiamo notizie come quella apparsa ieri di un Comune del Nord che ha deciso di incentivare i vigili che arrestano clandestini, istituendo così una vera e propria taglia. Giustamente il sindacato ha inviato un esposto alla prefettura per istigazione all'odio razziale mentre, secondo il sindaco, non ci sarebbe nulla di razzista in questa caccia allo straniero. Ecco allora che un provvedimento che voglia governare i flussi migratori, con l'intento di abolire il fenomeno della clandestinità e delle conseguenti forme di vero e proprio schiavismo, non potrà non essere accompagnato da una vigorosa attenzione a che tutte le forme di illegalità commesse a danno degli immigrati vengano energicamente combattute. L'impegno che deriverà dal nuovo provvedimento dovrà inoltre andare di pari passo con un'azione culturale e sociale di accoglienza e di integrazione. Esistono già, grazie all'impegno di molte meritevoli associazioni, esperienze preziose in questa direzione. Dovremo saperle aiutare e diffondere adeguatamente, in modo che tante speranze e progetti di vita possano trasformarsi in un arricchimento della nostra società, anziché essere respinte o in alcuni casi gettate per disperazione nelle mani sempre pronte della malavita.

Signor Presidente, vorrei fare innanzitutto un richiamo al principio di realtà, perché quello che stiamo svolgendo in quest'Aula non è un dibattito accademico.

Schematicamente - il tempo non consente gli approfondimenti che il tema richiederebbe - possiamo dire, senza tema di smentita e con tutto il rispetto nei confronti di queste politiche e di queste tradizioni culturali, che negli ultimi anni sono entrate in crisi e sono state drammaticamente smentite dai

Gran Bretagna, e quella laicista che è stata invece praticata soprattutto in Francia. La prima via puntava a un modello di integrazione al cui centro vi fossero le comunità

necessaria affinché l'immigrato diventasse cittadino. Era questa la tradizione del grande istitutore laico, l'*instituteur* francese, il custode delle tavole della cittadinanza che aveva il compito di trasferire di generazione in generazione. Signor Presidente, colleghi senatori, noi stiamo assistendo al fallimento di queste due vie ed è un fallimento confessato dagli stessi protagonisti di tali politiche.

Trevor Phillips, presidente della *Commission for racial equality* del Regno Unito, venne in Italia a dirci, a proposito del modello multiculturale: stiamo camminando a occhi chiusi verso il baratro e non abbiamo la forza di fermarci. Cosa fosse quel baratro lo abbiamo capito poco tempo dopo.

propose una revisione sostanziale di quella filosofia dell'integrazione che si era affermata anche attraverso la cosiddetta legge Stasi. È per questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che *leader* politici,

stanno revisionando profondamente le loro politiche, dando una stretta di vite alle politiche di immigrazione che avevano caratterizzato i loro programmi di Governo. Vede, signor Presidente, abbiamo apprezzato, più che i contenuti, i toni di alcuni interventi dei colleghi della maggioranza. Sappiamo perfettamente - lo diciamo anche ai signori del Governo - che l'immigrazione può essere una risorsa importante. Nessuno intende demonizzare il fenomeno. È troppo serio perché si compia demagogia su di esso. Ma sappiamo anche, per quel principio di realtà al quale prima mi appellavo,

decreto flussi si è trasformato, di fatto, in una sanatoria. Se su 520.000 domande presentate ne vengono accolte 520.000, quel provvedimento, colleghi della maggioranza, potete chiamarlo con i nomi più fantasiosi, anche «Bartolomeo» o «Filippo», ma tutti cittadini italiani capiranno che si tratta di una sanatoria di fatto. E poi, una legge sul ricongiungimento, che non considera i problemi enormi, ad esempio, legati alla condizione della donna immigrata, anche anche presenti nelle politiche di ricongiungimento, che molto spesso peggiorano la condizione di dipendenza della donna immigrata nel nostro Paese. Signor Presidente, mi permetta di dire a questo proposito che la polemica

dal Governo una politica sulla cittadinanza che si pone solamente un problema «quantitativo»: diminuire il numero degli anni per i quali è necessario

le risposte alle emergenze possono di fatto - questo è il vero rischio che tutti noi stiamo correndo - annullare la possibilità di elaborare una politica originale.

lassismo, da una parte, e xenofobia, dall'altra. Abbiamo già visto questa dinamica nella libertaria Olanda e non vogliamo che si ripeta anche in Italia. Per tali

Signor Presidente, la Presidenza ha chiesto un quarto d'ora di sospensione. Per quanto irrituale durante l'esame di una mozione, l'Aula ha assentito a tale richiesta. Mi permetto però di osservare che il quarto d'ora ha poi superato la mezz'ora. Questo non è accettabile

Signor Presidente, l'impianto delle due mozioni, sia per la sua ampiezza, che per il carattere di generalità degli impegni che propone, richiede doverosamente una premessa che riguarda l'essenza stessa...

Come dicevo, tale premessa doverosa riguarda l'essenza stessa delle politiche che il Governo intende promuovere e condurre in materia di immigrazione. Sento la necessità di fare questo anche in relazione e nel rispetto del dibattito svoltosi in quest'Aula, che ha portato all'attenzione della stessa alcune riflessioni

del fenomeno dell'immigrazione e alla luce di ciò il Governo stesso ha valutato le peculiarità e i limiti della legislazione vigente e anche la sua inidoneità a consentire un governo efficace e realistico di un fenomeno che ha dimensioni epocali. Nella primavera scorsa, il Segretario generale dell'ONU, presentando il dialogo ad alto livello su immigrazione e sviluppo, citava un dato che considero straordinario e che giudico sia sempre necessario avere a mente, quando si parla dell'immigrazione: Kofi Annan ivi riferiva che nel 2005 le persone che hanno lasciato il loro Paese di origine per recarsi a vivere e a lavorare in un'altra terra sono diventate 191 milioni

Credo che sia vero e importante riconoscere che rispetto a tale fenomeno il nostro dovere è di predisporre politiche di Governo. È stato detto da qualcuno, non per difenderci: esattamente, non per difenderci, ma per governare il fenomeno e indirizzarlo in una prospettiva di convivenza possibile, di coesistenza e di incontro tra tutti i caratteri che il fenomeno porta con sé e tra le stesse persone. L'attuale impianto normativo, a giudizio di questo Governo, si proponeva di fronteggiare l'immigrazione clandestina all'insegna di un maggior rigore, ma di fatto ha introdotto istituiti e disposizioni che alla prova dei fatti qualche volta si sono rivelati irrealistici, qualche altra volta inattuabili o inefficaci.

alla garanzia di un'occupazione, si è voluto, ad esempio, con quelle disposizioni (la cosiddetta legge Bossi-Fini), collegare l'ingresso sul territorio nazionale all'esistenza di un contratto di lavoro; ma per far questo si è dato vita ad un istituto, quello del contratto di soggiorno, che alla fine si è tradotto in periodiche regolarizzazioni e ha finito per favorire quell'immigrazione illegale che si proponeva di contrastare. Questo perché il modo in cui regola l'assunzione all'estero non è realistico, soprattutto per il personale non qualificato: nessuna famiglia assume una *baby-sitter*, affida i suoi affetti più cari, un anziano, un bambino ad una persona che non ha prima conosciuto. Inoltre, l'aver rigidamente legato la validità del permesso di soggiorno alla durata del contratto di lavoro, in presenza di un gran numero di contratti a termine di breve o brevissima durata, in un sistema statale che legifera sulla flessibilità quando non anche sulla precarietà del posto di lavoro, ha finito col produrre inefficienze sia per l'immigrato che per il datore di lavoro, favorendo il passaggio alla clandestinità degli immigrati che perdono il lavoro e ponendo problematiche molto delicate nella gestione dei cosiddetti *over stayer*. Allo stesso modo, si è approntato, sulla carta, un meccanismo delle espulsioni molto severo, ma che nei fatti si è rilevato poco efficace, perché non ha risolto i nodi esistenti sopratutto in tema di identificazione. Infine, per restare soltanto ai più macroscopici limiti dell'attuale sistema, si è voluta disegnare una normativa che sembra non tenere conto, ed anzi rifiutare, la portata storica del fenomeno dell'immigrazione dal Sud del mondo; quel fenomeno che lo stesso senatore Pisanu, quando era ministro dell'interno, indicò come un fenomeno che stava ponendo con forza all'attenzione dei suoi colleghi, degli allora Ministri. Si è data l'impressione di dimenticare che la forte pressione immigratoria di questi anni non pone soltanto problemi, ma offre anche delle opportunità. L'immigrazione sta cambiando il tessuto sociale dei Paesi di destinazione, ma anche dei Paesi di origine. In una Paese a bassa natalità come l'Italia, l'immigrazione garantisce la necessaria vitalità demografica - lo ricordava il senatore Livi Bacci - e contribuisce alla sostenibilità del sistema pensionistico; i lavoratori immigrati sono una risorsa fondamentale per le nostre imprese e le nostre famiglie e tutte le analisi economiche concordano sul fatto che l'immigrazione produce sviluppo e non toglie lavoro ai residenti; che un'immigrazione regolare riduce fortemente il tasso di delittuosità tra gli immigrati; che l'immigrazione di alto livello professionale, in particolare, è uno strumento essenziale di competitività. Il fenomeno dell'immigrazione è in costante evoluzione e richiede un dinamismo normativo che non può fermarsi ad una mera difesa di principio della legislazione vigente. Proprio su questo la Caritas, che ieri ha presentato il proprio rapporto annuale sull'immigrazione, ha invitato le forze politiche ad andare al di là dell'alternanza, a considerare che quello dell'immigrazione è un tema che va affrontato fuori delle strumentalizzazioni politiche, cioè fuori dalla necessità politica di voler rigettare sull'altra parte le responsabilità e fuori - direi - anche della volontà di strumentalizzare le paure e l'inquietudine presenti tra i cittadini. Queste riflessioni hanno indotto il Governo a maturare il convincimento che vi siano aspetti della materia su cui un intervento correttivo non è più rinviabile. E questo occorre farlo soprattutto in relazione all'obiettivo di favorire l'immigrazione regolare nel nostro Paese e quindi rendere questa un'immigrazione che dia un'opportunità alle persone che vengono a vivere e a lavorare tra noi.

vigente. Il fatto che il 14 marzo 2006 agli sportelli postali siano giunte 481.105 domande non è una responsabilità imputabile a questo Governo. È un dato di realtà che tutti abbiamo il dovere di guardare e che abbiamo voluto guardare ascoltando le associazioni datoriali che ci dicevano che quella domanda rispondeva ad un'esigenza occupazionale effettiva, che doveva essere presa in considerazione. Da qui, in conformità con la legge Bossi-Fini, è nata l'idea di presentare al Paese un secondo decreto flussi; decreto che la legislazione attuale consente al Governo di adottare.

non si parlasse impropriamente (come è stato fatto, non dal Governo, non dalla maggioranza, ma dall'opposizione) di una sanatoria perché di sanatoria non si tratta, a meno che non si voglia chiamare sanatoria anche quella operata dal Governo precedente ed avvenuta ai sensi di legge.

si è inteso intraprendere un percorso che consenta di individuare quegli strumenti normativi che sanzionino i comportamenti illegali degli immigrati e soprattutto di chi favorisce

per quanto riguarda la mozione unitaria presentata dall'opposizione sottolineo con serenità che vi sono aspetti, soprattutto nella parte di premessa, che non sono assolutamente condivisibili e non appartengono alla politica del Governo.

poiché si trovano compresi in una mozione che prevalentemente ha istanze non condivisibili, il parere del Governo è contrario alla una nuova finestra"). Vorrei comunicare all'Assemblea che è presente in tribuna il ministro della giustizia della Repubblica di Capo Verde, Manuel Andrade, accompagnato da una delegazione guidata dall'ambasciatore presso la Repubblica italiana, dottor José

una mozione che si impegna sul nuovo e che tenta strade nuove, accogliendo il parere di persone di buona volontà e, se vogliamo far riferimento alle considerazioni più volte espresse dal ministro Amato,

D'altra parte, il senatore Quagliariello ci ha invitato a svolgere alcune riflessioni molto condivisibili di sistema sulla difficoltà dell'Europa a gestire ipotesi anche diverse di governo delle migrazioni. È uscito da poco un bellissimo libro «Goodbye, Europa», degli economisti Alesina e Giavazzi, in cui vi è un capitolo molto interessante e recentissimo dedicato proprio alle ultime analisi dei flussi migratori e dei relativi dati. Chi vorrà misurarsi con il pensiero di questi economisti liberali sul governo dei flussi migratori vedrà e potrà esaminare come

tecnici e scientifici che dai Paesi dell'Est fra quattro-cinque anni si proporranno nell'Europa occidentale a seguito del libero mercato delle migrazioni, consenta processi di integrazione e di realistico governo della questione: un'integrazione problematica ma fattiva. Questo dicono economisti liberali, a cui dovrebbe andare l'attenzione vigile anche di parte della nostra opposizione. Per quanto riguarda i provvedimenti che in questa sede sono stati illustrati, ho avuto modo di dare un'occhiata rapida alla mozione unificata presentata dall'opposizione. Fate bene, colleghi dell'opposizione, a parlare di Nazione ombra,

di tanti talenti, io credo - e penso che anche voi potreste convenire - abbia bisogno di strumenti più raffinati, processuali e misurati in avanti. Voi stessi dovreste chiedervi perché non ha funzionato il contratto di soggiorno, perché è sempre stato aggirato, perché prima si viene in Italia e poi

pace, integrazione, come si vede nelle famiglie immigrate a Torino, a Padova, a Roma. Io vengo da Torino, conosco benissimo com'è stata l'evoluzione, ad esempio, di zone critiche come San Salvario. La politica dei ricongiungimenti oculati aiuta (e giustamente; ne parlate anche voi) a risolvere il problema enorme dell'integrazione delle donne di cultura islamica; si può, grazie ad un'oculata politica dei ricongiungimenti, trovare una cooperazione interessante e fervida di culture. quindi con reale convinzione la mozione della maggioranza, ripeto, perché è una mozione che sfida il nuovo e guarda al futuro.

colleghe e colleghi, signori del Governo, alla fine del 2004 i cittadini stranieri nei 25 Stati membri dell'Unione, escludendo quelli che hanno già acquisito la cittadinanza, sono risultati 26.061.000 26.061.000 su una popolazione di 457 milioni di abitanti. E un'incidenza di poco superiore al 5 per cento, con punte del 9 in Germania e in Austria, dell'8 in Spagna, del 5 nel Regno Unito e in Francia e del 4 per cento in Italia. L'Unione Europea si presenta così come un'area ad alta concentrazione di immigrati, la cui presenza costituisce una necessità demografica perché il vecchio continente, anche se è prevista un'immigrazione netta di 40 milioni di persone nel 2050, vedrà comunque diminuire di 7 milioni di unità la popolazione nel suo complesso e di 52 milioni di unità la popolazione in età da lavoro. Nonostante queste implicazioni quantitative e la lunga esperienza storica per essere stata una grande area di esodo fino alla Seconda guerra mondiale, l'Unione Europea sta vivendo un atteggiamento tormentato nei confronti dell'immigrazione. È costitutiva dell'idea dell'Europa unita la libertà di viaggiare e di lavorare, ma essa si intreccia, è connessa con la paura dell'invasione, della sottrazione, del *dumping* sociale. In Italia l'immigrazione diventerà sempre più l'unico fattore di crescita demografica; gli immigrati sono in Italia una popolazione giovane, concentrata per il 70 per cento nelle fasce di età dai 15 ai 44 anni. Sul piano del lavoro, lo stesso Franco Frattini, vice presidente della Commissione europea, ha preso atto che l'Italia, come tutta l'Europa, ha bisogno di manodopera straniera; il rispetto delle leggi deve essere - egli dice - coniugato con la solidarietà. però, è solo una parte, Presidente: è la cornice entro cui poniamo la tela che è ben più fitta ed intrecciata delle questioni che riguardano l'immigrazione.

fame e violenza. Siamo in Europa ad un tornante storico che rimette a tema anche la costruzione del modello di rapporto tra europei, indigeni e migranti. Su questa strada non vi sono scorciatoie di natura repressiva, né integrazione forzata che non riconosca le diversità culturali e religiose degli altri. E non si pensi sempre che il proprio modello sia il migliore. Su questa strada vanno ricostruiti i paradigmi dell'accoglienza, della solidarietà e dei diritti. Il provvedimento sui flussi, avanzato dal ministro Ferrero, altro non è che un provvedimento di buonsenso, che consentirebbe di integrare con 350.000 lavoratori la quota di ingressi per lavoro che avevamo programmato il 15 febbraio. Riteniamo che la scelta di riaprire i flussi d'ingresso adeguandoli all'entità delle domande di nulla osta presentate in occasione del primo decreto flussi

per nostra responsabilità. La grande maggioranza di domande di nulla osta riguarda lavoratori non comunitari già presenti nel nostro Paese e in attesa di regolarizzazione della propria situazione lavorativa e di soggiorno. Si tratta dunque di una situazione drammatica che penalizza oltre ai lavoratori e le lavoratrici non comunitari, anche i datori di lavoro e rivela con assoluta chiarezza i profondi limiti ed incongruenze che caratterizzano i dispositivi attualmente preposti alla regolamentazione degli ingressi per lavoro nel nostro Paese. Paese. Insomma, siamo di fronte ad una grande questione democratica, a cui non si può rispondere con uno «stato penale globale», come dice Eligio Resta. No, non si può non si può introdurre un diritto differente per i migranti, né si può risolvere il problema con la farraginosità di una legge tuttora in vigore; bisogna rispondere al bisogno di sicurezza con la certezza del diritto per tutte e per tutti e non abbiamo neppure ancora - è per questo che lo chiediamo nella nostra mozione - ratificato la convenzione dell'ONU sui diritti dei migranti e delle loro famiglie. Non potremmo votare la mozione presentata dal centro-destra, che vede come

lasciare la propria terra, non è facile rompere quel legame. Vi siete mai chiesti perché mai il marocchino, che è avvolto la sera nei cartoni e forse pensa e sogna i propri cieli africani, è qui da noi? Vi siete posti il problema, forse, che il modo di vedere l'economia che ha trovato nelle guerre il proprio strumento sia la causa di questo? Credo allora che davvero non potremmo votare quella mozione e quindi votiamo la nostra, perché l'altra non comprende e non vuole comprendere che le ragioni di questi flussi migratori, di questi spostamenti di popoli sono qui da noi, sono nell'Occidente, che in qualche modo produce devastazione e sfruttamento. Discuteremo anche dell'Africa, signor Presidente e allora scopriremo come quel popolo, quando riusciremo a parlarne, oggi forse potrebbe dire di sé che è stato davvero un popolo del tutto depredato. *(Applausi

esaustiva. In effetti quello che ci ha detto la rappresentante del Governo che è intervenuta oggi, anche se con una certa limitazione temporale che impediva di svolgere compiutamente un discorso così importante, è altrettanto chiarificatore rispetto a quanto è scritto nelle mozioni che sono state presentate e che sono oggetto del nostro voto. Sono un po' preoccupato perché, a questo punto, se speravamo di avere, oltre al dibattito parlamentare, delle risposte sulla politica dell'immigrazione da parte del Governo, abbiamo ottenuto delle risposte che da un lato

di Paesi della costa sud-mediterranea (come è stato anche fatto in passato) per evitare che ci siano i viaggi della morte e lo sfruttamento schiavista da parte degli scafisti. Alla luce di queste sue affermazioni, favorevoli di principio, non esistono però delle proposte concrete di controllo dei flussi migratori. Non vorrei che, a quanto ho sentito dai colleghi poco fa, passasse l'idea molto pericolosa e che sta ingenerando

in base alla necessità. Credo che questa sia un'espressione assolutamente pericolosa, da un lato, perché porterebbe ovviamente alla teorica assunzione di tutto il mondo immigrato che volesse entrare in Italia - ed è questa la direzione verso cui si va - e, dall'altro, perché ingenera comunque delle speranze che danno

causa della recrudescenza degli sbarchi dei clandestini nel nostro Paese. Io avrei allora avuto il piacere, oltre ad ascoltare enunciazioni di principio, di sapere quali tipi di azioni diplomatiche forti volete compiere nei confronti di un Paese che si sta dimostrando strumento conscio conscio (che non subisce quindi flussi che vengono da chissà dove) in questo trasbordo di disgraziati, purtroppo sfruttati, dalla costa dell'Africa all'Italia. Le sue risposte, signor Sottosegretario,

dell'acquisizione della cittadinanza da parte di minori, prevede che a dare il consenso per la patria potestà sia il genitore che, secondo la legislazione del Paese d'origine, gode della patria potestà.

del centro-destra con un'unica mozione comune e si è preoccupato anche di aprire questa mozione, inserendo elementi che potessero facilitare un giudizio positivo da parte del Governo. L'Esecutivo ha rilevato l'esistenza di questi elementi, ma il giudizio positivo non lo ha dato. A mio parere, il Governo sbaglia, sbaglia per due motivi: il primo è che è in atto nella maggioranza un dibattito. Ci sono quelli che puntano ad una autosufficienza blindata, perché hanno la sensazione che se si apre davvero un dialogo in quest'Aula molte posizioni ideologiche presenti nella maggioranza si scioglieranno e verranno restituite a quella posizione minoritaria minoritaria e marginale che hanno, effettivamente, nella vita del Paese. Si tratta di un errore, perché non vi dirò che non avete la maggioranza in quest'Aula, l'avete, ma è una maggioranza precaria, esposta ad ogni soffio di vento. Sarebbe nel vostro interesse avere il pieno rispetto della funzione del Parlamento e l'atteggiamento, che è comune nei Parlamenti europei, della ricerca di tutte le convergenze possibili, valorizzando il contributo dell'opposizione. Non avete voluto cogliere questa occasione. Il secondo motivo per cui questo è un errore è che la questione dell'immigrazione dell'immigrazione è troppo importante per affrontarla con delle retoriche di parte; è una tematica che mette in gioco il futuro del pianeta, ma anche il futuro di questa Nazione, dell'identità nazionale italiana. Per noi, infatti, non è irrilevante sapere se fra cinquanta anni ci saranno ancora gli italiani in Italia, se si parlerà ancora questa lingua o se se ne parlerà un'altra, se i riferimenti di Dante, di Michelangelo, di Petrarca saranno ancora quelli traenti per un'identità nazionale italiana. Ogni popolo ha diritto ad un'identità, ogni terra è legata ad una cultura. Questa terra è legata ad una cultura umanistica e cristiana; non lo dice l'ex ministro bigotto Buttiglione, ma il laicissimo Carlo Azeglio Ciampi nel suo discorso per la consegna del «Premio Carlo Magno». Siamo preoccupati per questa identità e ricordiamo che l'immigrato è una persona umana. Non possiamo pensare di importare braccia, si importano uomini che hanno diritti e che devono assumere doveri: hanno diritto al rispetto della loro cultura, devono assumere il dovere di rispettare la nostra cultura. Non si importano solo braccia, perché l'uomo è dentro un tessuto di rapporti affettivi e sociali. Bene i ricongiungimenti; certo, la presenza delle donne modera qualunque comunità ed è un fattore fondamentale di integrazione, ma attenti al modo in cui si fanno i ricongiungimenti, perché, signor Sottosegretario, esiste un patrimonio di istituzioni, di fondi, di beni che sono destinati all'assistenza dei poveri in Italia.

con i Paesi rivieraschi per stringere con loro accordi di cooperazione e sviluppo, chiedendo in cambio sostegno per il controllo dell'immigrazione clandestina. Di questa conferenza non si parla più.

La politica europea in questo ambito è ferma. Si potrebbe, a legislazione vigente, realizzare la comunitarizzazione di buona parte delle competenze in questa materia anche senza una nuova Costituzione.

poi il tema della formazione di una collaborazione per definire lo *status* di rifugiato. Lì qualcosa è stato intrapreso, ma molto lentamente. Concludo

con l'onorevole Mantovano, anche perché credo che abbiamo già dato abbondantemente negli anni scorsi da questo punto di vista. Vorrei però leggere all'Aula un annuncio del signor Richard Baucher,

e il 1976 ben 26 milioni di espatri) sarebbe stato sottoposto a riesame, insieme all'Uruguay, alla Slovenia, all'Argentina e ad altri, in merito alla possibilità, per i suoi cittadini, di entrare negli Stati Uniti senza visto. Il motivo di tale decisione scaturisce dalla convinzione dell'INS (Servizio immigrazione e naturalizzazione) che una parte significativa dell'imponente mole di ingressi di italiani (circa 800.000 unità in quegli anni) vada configurata come immigrazione clandestina. Molti nostri connazionali, cioè, utilizzerebbero il visto turistico per risiedere clandestinamente in America ben oltre i novanta giorni previsti dalla legge. Secondo la CNN buona parte di clandestini italiani sarebbe costituita da musicisti, girovaghi, pizzaioli abusivi e - ahimè! - manovalanza mafiosa.

che sappia tenere conto della contemporaneità, quindi di che cosa sta accadendo all'interno del pianeta. È altrettanto evidente che la cosiddetta guerra globale permanente non fa altro che creare ulteriori disagi

metallo del disonore, ossia malattie legate all'uranio impoverito o alle nanoparticelle, come risulta dagli ultimi studi effettuati. Ebbene, provate a pensare in quali condizioni vengono lasciati quei territori.

che la sfera dei diritti sia un vero e proprio ammortizzatore sociale rispetto ai conflitti esistenti all'interno della nostra società. Quindi è necessaria una legge certa sul dritto di cittadinanza, che non divida più le persone in cittadini di serie A e cittadini di serie B, come ad esempio è stato fatto dalla legge Bossi-Fini. Non si capisce perché, per un reato di tipo amministrativo, persone che vengono da altri Paesi, magari di altre religioni e possibilmente anche di altro colore, siano costrette a forme di privazione della libertà di tipo carcerario, magari privatizzate, cosa che non esiste per noi all'interno di questo territorio. Questo è un altro dei temi da trattare. Quindi, più diritti (mi rivolgo al Sottosegretario perché so che stiamo andando in questa direzione, come deciso tra l'altro al tavolo dell'Unione sull'immigrazione quando preparammo il programma); più diritti, non vivendo gli immigrati solo e unicamente come forza lavoro: sono persone ed è su questo probabilmente che dobbiamo tentare di costruire di costruire le nostre politiche sul tema dell'immigrazione. Come Verdi, a quel tavolo avevamo proposto la creazione del Ministero dell'immigrazione, perché riteniamo che oggi voler governare il tema dei flussi migratori richieda un vero e proprio Ministero che sappia affrontare a 360 gradi il tema dell'immigrazione, che sta diventando una sorta di leva rispetto

sui diritti, sul diritto al voto e quant'altro proprio perché l'immigrazione ci avvolge a 360 gradi. Su questo credo dovremo trovare delle risposte.

è vincolare il Governo, con il voto del Parlamento, a seguire, in materia di immigrazione, una politica conforme agli orientamenti dell'Unione Europea, ma vorrei dire in generale una politica *tout* perché se è legittimo che maggioranza e Governo propongano una disciplina dell'immigrazione diversa rispetto a quella introdotta dalla maggioranza precedente, è un fatto che nei suoi cinque mesi e otto giorni di vita il Governo Prodi non ha depositato nessun disegno di legge organico e alternativo alla legge in vigore, per permettere il confronto tra prospettive diverse su un tema così cruciale. Da questo punto di vista ha ragione il senatore Bulgarelli a lamentarsene. Esiste un motivo per tutto questo. Ciò è accaduto, infatti, esclusivamente per i gravi contrasti interni al Governo e alla maggioranza, perché ad un ministro Ferrero che propone di dare il permesso di soggiorno al clandestino che denuncia il datore di lavoro che lo impiega in nero si contrappone un ministro Amato che definisce questa proposta il più grande regalo che si può fare alla criminalità organizzata. In realtà, il ministro Amato ha illustrato come immagina di modificare l'attuale disciplina sull'immigrazione: per esempio con ingressi privilegiati di lavoratori altamente qualificati (peccato che questo sia già contenuto nel testo della Fini-Bossi, all'articolo 27 per esempio con i corsi di formazione nei Paesi di origine (ma anche questo si trova all'articolo 23 dello stesso decreto legislativo); per esempio con la distinzione tra Centri di permanenza temporanea e centri di prima accoglienza (questo non solo è scritto nella legge, ma anche concretamente attuato); per esempio con la programmazione triennale e così via. Se il ministro Amato lo ritiene, visto che condivide a tal punto la normativa in vigore, potremmo accogliere la sua firma in calce alla Fini-Bossi e chiamarla Fini-Bossi-Amato. Se la maggioranza non raggiunge, al proprio interno, un accordo, il Governo prova ad aggirare l'attuale disciplina con una serie frammentata di atti amministrativi, il decreto flussi integrativo, o di singole norme inserite in testi che trattano tutt'altro; non ne faccio l'elenco, che è contenuto nella mozione a firma mia e dei colleghi di Alleanza Nazionale. Vorrei dire alla sottosegretario Lucidi che noi siamo sempre disponibili a soluzioni concrete su singoli punti. Il problema è che voi state sovvertendo in maniera indiretta l'intero sistemo senza affrontare direttamente la sua discussione e, poiché seguiamo poiché seguiamo tutti i siti Internet, sappiamo anche che la criminalità organizzata, quella che sfrutta l'immigrazione clandestina, è in grado di dare indicazioni sul dove andare e sul come farlo. Proprio oggi la stampa quotidiana informa con dovizia di particolari sul punto. Le istruzioni seguono e cercano di adattarsi alle modifiche delle norme e delle politiche di Governo. Da fine maggio, grazie ai vostri annunci, le istruzioni sono semplicissime: clandestini di tutto il mondo, non «unitevi», ma «andate in Italia».

mentre la Spagna prospetta l'espulsione di 800.000 clandestini e blinda Ceuta e Melilla - sto parlano di due Stati europei con Governi di sinistra - ... *(Brusìo)*.

sanare la propria posizione, come ha fatto il decreto flussi integrativo che - lo ribadisco al rappresentante del Governo, che parla al telefono - è una sanatoria illegale e illecita; è possibile allargare la propria presenza con l'estensione, nei termini amplissimi che si vogliono introdurre, dei ricongiungimenti familiari. Tutto questo senza rischi di espulsione, perché il Governo sta riducendo i posti nei CPT; rinuncia a rimandare nei Paesi d'origine addirittura quei clandestini che sono stati condannati e poi scarcerati grazie al vostro indulto e, dopo cinque anni, tutti cittadini!

non dovete utilizzare il dato del 2006 se non a partire da quello sciagurato giorno - il 18 maggio di quest'anno - in cui avete iniziato a «sgovernare». Paragonando questo bimestre,

Quello che accade in Europa ha incidenza sull'Italia, perché, mentre poco più di un anno fa i marocchini che arrivavano clandestinamente a Lampedusa erano il 4 per cento, adesso sono il 40 per cento. In Puglia sono ripresi gli sbarchi. L'ultimo sbarco risaliva all'agosto del 2002. Quattro anni di blocco; nell'agosto del 2006 Internet arriva anche nei Paesi da cui è più facile arrivare in Puglia. Concludo, signor Presidente, dicendo che in realtà l'immigrazione è uno dei terreni privilegiati sui quali pesa in modo determinante la pregiudiziale ideologica della sinistra radicale

pur di ossequiare questa pregiudiziale ideologica. Ho annotato infatti, persino nelle parole, ciò che ha detto in discussione generale il senatore Rossi Fernando quando è arrivato a chiedere il ricongiungimento familiare con due mogli, in ossequio al rispetto delle regole di inciviltà che vigono in altri Paesi. Alla faccia del riconoscimento delle eguali dignità tra uomo e donna che la sinistra vorrebbe insegnarci quotidianamente! La sinistra radicale fa tutto questo con fini dichiarati di lucro (elettorale, ovviamente, non oso dire altro), come ha detto, con estrema chiarezza, il ministro Ferrero sulle colonne del «Corriere della Sera» lo scorso mese di agosto. Secondo il Ministro, da questo meccanismo, sanatoria

la vostra politica sull'immigrazione non è solo a favore dei clandestini e di chi li sfrutta; ponendo l'Italia fuori dall'Europa, è una politica clandestina di un Governo ormai clandestino che proprio per questo va espulso insieme con i clandestini.

Forza Italia voterà a favore della mozione unificata presentata dall'opposizione che affronta la scellerata politica del Governo sul tema dell'immigrazione. Voterà quindi contro la mozione presentata chiediamoci: qual è stata la risposta politica dell'attuale Governo di fronte alle continue emergenze dell'immigrazione? È amaro constatare che a livello locale, in una città importante come Padova, la soluzione è stata vista nella costruzione di un muro che è l'emblema del fallimento, dell'incapacità di garantire la legalità

si dice che dobbiamo dominare il fenomeno dell'immigrazione attraverso accordi internazionali con i Paesi dai quali gli immigrati provengono, con politiche europee di contenimento,

il che comporta un problema delicato e grave allo stesso tempo: la legittimazione dell'esistente da parte dello Stato, cioè la legittimazione della clandestinità. Il tutto senza chiedersi come si affronti il rapporto dialettico tra immigrazione e integrazione, né quale impatto potrà avere un'immigrazione massiccia

né un problema di anni per la cittadinanza: ridurre a questo la discussione mi pare banale. Il problema è capire come gli immigrati si possano inserire nella nostra società. A tale proposito, vorrei ricordare di Hina**,** di Elena Lonati, di tanti casi simili successi in Europa. Il ministro Amato aveva detto che sarebbero stati bloccati i flussi migratori fino a che non si fosse realizzata quella società integrata, che prevede il rispetto dei diritti e della dignità della donna e, quindi, i princìpi della nostra società. Si sono risolti questi problemi? Non credo se è scoppiata proprio in questi giorni la questione del velo, il simbolo di una limitazione della libertà delle donne, di una volontà di non integrazione. Allora, non possiamo applicare la facile equazione «immigrazione facile uguale integrazione immediata». Gli sbarchi clandestini, Elena Lonati, Hina, via Anelli di Padova, il velo sono fatti che dimostrano e che stanno a ricordarci che i problemi non si risolvono dietro un muro di latta, né nascondendo la polvere sotto il tappeto. I cittadini richiedono a grande voce sicurezza e legalità. È una preoccupazione emersa in maniera quasi prepotente anche nei sondaggi recenti e la politica scellerata di questo Governo va in direzione esattamente contraria: è contro la legalità, è contro la sicurezza dei cittadini ed è anche contro la tanto sbandierata solidarietà. Non si può invocare la solidarietà senza fornire, come aveva fatto la legge Bossi-fini, casa e lavoro, senza garantire quella dignità, che è il presupposto di ogni umana esistenza.

Presidente, spero di fare cosa gradita all'Assemblea, parlando soltanto un minuto e consegnando

Mantovano. So bene quale è l'importanza dei decreti sui flussi migratori e so bene qual è il rilievo che ha il buon funzionamento dei centri dei centri di accoglienza. Sono questioni molto importanti. Siamo tutti tenuti a seguirle con molta attenzione. Ma lei crede veramente che agli inizi del terzo millennio, in un mondo globalizzato, con una mobilità sostenuta come la nostra, siano poi le misure amministrative di un solo Stato, di una sola Nazione, di un solo Paese a poter non dico fermare, ma anche solo rallentare rallentare l'andamento dei flussi migratori? Lei non pensa che ci troviamo davanti ad un fenomeno di portata epocale, che può essere controllato soltanto con politiche internazionali nei confronti del Terzo e del Quarto mondo? Allora le chiedo questo, senatore Mantovano: l'Italia negli ultimi sei anni ha rimesso debiti nei confronti dell'Africa, dei Paesi del Quarto mondo per due miliardi e mezzo. il Governo, presieduto dal presidente Berlusconi, anche in modo consistente quando nel 2001, in occasione del G8, fece venire in Italia i Capi di sei Governi africani e diede inizio ad una stagione di nuovi rapporti con il continente africano. Il Governo Prodi ha raddoppiato nella finanziaria 2007 il contributo per la cooperazione. Le chiedo, senatore Mantovano, per quale motivo la sua mozione conteneva nelle premesse - come ha ricordato il rappresentante del Governo - considerazioni politiche che hanno reso impossibile qualsiasi contatto tra noi e qualsiasi possibilità di

faccio riferimento alle norme del nostro Regolamento che riguardano le modalità di votazione. Apprezzo la sua fatica, ma le chiedo di evitare che qui arrivino energumeni a minacciare i senatori.

Signor Presidente, vorrei proporre che, stando tutti seduti, un

Presidente, credo che oltre all'invito a stare seduti, risolverebbe tutti i problemi...

Non cominciamo adesso ad urlare,

della nostra Repubblica: il senatore Oscar Luigi Scalfaro, persona equilibrata, è stato accusato di complicità in un assassinio nel post-Liberazione, perché pare abbia commesso un errore giudiziario. Conoscendo la personalità assolutamente limpida del senatore Scalfaro, chiediamo che vi sia un giurì o una sua dichiarazione per sgombrare il campo da questo equivoco, perché pare sia stato complice di un errore giudiziario che ha portato alla fucilazione

Presidente, la questione dei voti doppi e tripli non può essere risolta, come giustamente lei ha fatto rilevare, nella maniera in cui si sta purtroppo risolvendo.

la panacea di tutti i mali, ma riduce il disdoro che tutti quanti noi riceviamo da simili situazioni, a prescindere da maggioranza e opposizione. Le chiederei, su tale questione, di fare qualche passo avanti. Il Gruppo dell'Ulivo sta aspettando dalla Presidenza la comunicazione di quali sono i posti

è possibile richiedere che il voto elettronico non avvenga solo, come si sta facendo, con il sistema fisso (nel senso che è sufficiente premere il pulsante e il voto rimane), ma è possibile chiedere anche il voto con la compressione del tasto permanente. Il voto cioè non rimane: bisogna premere il tasto e tenere la mano ferma; il che, signor Presidente, comporterebbe...

hanno adottato sistemi di votazione con l'impronta digitale che eviterebbero ogni e qualsiasi possibilità di confusione. E' una questione che non riguarda né la maggioranza né l'opposizione - chi è senza peccato scagli la prima pietra - però, signor Presidente, penso che nell'interesse dell'Istituzione una qualche soluzione debba essere trovata.

che la citazione evangelica dovrebbe essere non «chi è senza peccato», ma «chi è senza il peccato». La notazione configura una diversità assoluta nella storiografia evangelica e di questo, se vuole, potremo anche parlare dopo. Il punto principale di cui all'intervento sta nel fatto che ho sentito più volte - certamente non sono uno dei senatori più anziani in quest'Aula, ma neanche uno dei più giovani, e sono stato brevemente anche alla Camera dei deputati - la continua volontà, da parte di chi è stato invece molto tempo alla Camera dei deputati, di riportarne in questa

fare esternazioni o proposte che non hanno un fondamento, ancorché giuridico, di prassi, di volontà, di capacità, di possibilità, dovremmo fare un ragionamento un po' più serio. Non me ne voglia il senatore Boccia, ma le sue

invece nella serietà, nella capacità, nella preparazione; in tutt'altri aspetti, quindi, che non nel meccanismo del voto, nella tessera, nell'assenza o nel gridare l'un contro l'altro in maniera scalmanata, come ogni tanto avviene in quest'Aula.

minoranza, al punto che applaude quando vince e ciò è sintomatico, perché di solito la notizia è quando vinciamo noi, non quando vince la maggioranza. Questa maggioranza, invece, applaude quando vince. Dica loro di star tranquilli, che ci sono i senatori segretari, che c'è un Presidente di cui si devono fidare ancora di più

Le assicuro, Presidente, che sarà l'ultima volta, perché non accetto provocazioni del genere. Oggi mi sono autocontrollato; se la prossima volta qualcuno verrà qui a fare delle provocazioni

elettorale varata prima delle elezioni, il risultato della composizione di quest'Aula proviene anche dal voto del popolo italiano.

la proposta avanzata dal mio amico Storace: quando vedrà una situazione che minaccia di andare verso l'uso della forza, lei, che deve essere abituato aver tenuto assemblee sindacali piuttosto vivaci, deve esercitare il suo potere, sospendere la seduta e, fino al momento in cui non si saranno verificate le condizioni giustamente da lei imposte, cioè che ognuno sia seduto al proprio posto, lei non deve riaprire la votazione.